"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

il relatore ha seguito l'intero dibattito che si è sviluppato ieri e ritiene di selezionare alcune delle questioni poste per poste per la importanza degli argomenti e anche per il modo equilibrato e completo con il quale sono state trattate. Ritengo di dare la precedenza alla questione che concerne quell'attribuzione di rilevanza

che l'aggettivo «rilevante», che compare nell'articolo 2621 e, parzialmente, nell'articolo 2622, porrebbe questioni di costituzionalità. Ovviamente, io non torno sulla questione di costituzionalità di natura pregiudiziale ma, siccome la questione è riproposta attraverso emendamenti volti a determinare la soppressione dell'attributo di rilevanza, ha carattere di attualità. Intanto, parto dalla più volte evocata sentenza n. 247 del 1989 della Corte costituzionale per segnalarne, per un verso, la scarsa utilizzabilità a questi fini e, per altro verso, per segnalare come essa non costituisca il termine di paragone, a livello di costituzionalità, dell'attributo «rilevante». Do conto della mia prima affermazione. La sentenza, ovviamente, pone un problema di costituzionalità con riferimento ad aggettivi ed ad attributi di natura quantitativa, ma indeterminati, nel solco di una ovvia giurisprudenza costituzionale che vuole che il limite tra il vietato e il consentito sia segnato in maniera certa dal legislatore e che, quindi, non si scarichi sul giudice la decisione la decisione di stabilire ciò che è reato rispetto a ciò che non lo è. Rispetto ad una tale sequenza farebbe ostacolo l'articolo 25, capoverso, della nostra Costituzione oltre che l'articolo 3 ma, soprattutto, il monopolio riconosciuto esclusivamente in capo al legislativo di stabilire ciò che può essere qualificato come reato ovvero no. no. Quella sentenza afferma un principio ben più complesso rispetto a quello che è stato, al contrario, rappresentato dei suoi contenuti. dice che non è possibile che l'intero carico di disvalore penalistico gravi su elementi indeterminati di natura quantitativa, dovendo, al contrario, ritenersi costituzionale una norma penale la quale si avvalga di elementi quantitativi, ancorché da determinarsi, ma che, con riferimento al disvalore di condotta, sia talmente ricca e pregnante e costituita da elementi che demarcano il consentito rispetto al vietato da risultare, già sul piano del disvalore della condotta, sufficientemente determinata. Ora, questa norma può essere accusata di tutto tranne che di indeterminatezza sul piano della condotta. Abbiamo una norma che si avvale dell'espressione «fatti», per di più «materiali e rilevanti» - vedremo poi cosa vuole dire l'attributo «rilevante» è costruita integralmente su una condotta artificiosa, concretamente idonea ad ingannare; per di più, sul versante della componente soggettiva del fatto, si avvale dell'avverbio «consapevolmente», di cui darò conto da qui a qualche minuto, ma che certamente completa il versante di determinatezza della condotta. condotta. Si tratta dunque di una norma semmai iperdeterminata dal punto di vista dei suoi elementi di struttura, dimostrativi di un disvalore di condotta, già sufficiente a determinarla. dicevo nella parte iniziale del mio intervento, paradossalmente il discorso fatto in ordine alla sentenza n. 247 del 1989 è del tutto inutile e superfluo, perché esso implica che l'espressione «rilevante» venga interpretata quale elemento quantitativo non numerico, dimostrativo di una certa soglia indeterminata, sempre di tipo quantitativo, che rimetterebbe al giudice il compito di determinare oltre quale livello quantitativo la condotta è punibile e, correlativamente, al di sotto di quale livello quantitativo essa non lo è. Dunque, il reclamo dell'efficacia, d'ostacolo della sentenza n. 247 del 1989, parte da un'interpretazione unilaterale dell'attributo «rilevante», assegnandogli per l'appunto - lo ripeto per l'ultima volta quella funzione di indicazione di dato quantitativo volto a discriminare il consentito dal penalmente rilevante. Le cose non stanno però assolutamente in questi termini

l'attributo di rilevanza si accompagna. Rilevante non è attributo di un sostantivo come «quantità», «misura» o «variazione» - ossia di un sostantivo dimostrativo, che già di per se stesso fa riferimento a dati quantitativi

nel solco di una giurisprudenza consolidata e certa della nostra Corte costituzionale in materia di principio di offensività, inteso non soltanto in senso astratto - ovvero la norma deve contenere elementi dimostrativi della capacità del fatto di offendere - ma anche in concreto, imponendo la Corte costituzionale non soltanto al legislatore di scrivere norme offensive, ma anche al giudice di interpretarle in aderenza, orientando la sua interpretazione al principio di offensività.

principio che si sposa perfettamente con il correlativo principio di offensività - si comprende come la norma sia organica: essa evoca la necessità di un fatto, impone che esso sia materiale ulteriormente, in terza battuta, impone che esso sia un fatto rilevante sul piano della sua capacità di offendere il bene giuridico. Questa espressione - che si può ritenere ritenere semmai enfatica, ripetitiva e ridondante, ma non inutile, nella misura in cui la norma deve chiarire ed evitare conflitti di interpretazione - si completa con l'espressione «concretamente idoneo ad indurre in errore»

si contrassegnano tutti per la necessità di dimostrare ulteriormente in concreto la capacità offensiva della condotta. ambiti dogmatici se ricordassi non soltanto il pensiero di illustri penalisti come Marcello Gallo, quindi dell'intera scuola di Torino, ma anche di altri illustri penalisti come Franco Bricola, che proprio sul sul terreno dei delitti di falso hanno ricostruito la teoria dell'offesa e la necessità di evitare che fatti formalmente conformi al tipo siano punibili, al contrario della necessità di individuare, all'interno della generalista categoria dei fatti conformi al tipo, solo quella meritevole di intervento penalistico, ossia dei fatti effettivamente e concretamente offensivi e tali da determinare in concreto quell'offesa che rende il fatto dotato di una sua reale pregnanza penalistica; e tra l'altro del tutto perfettamente conforme a Costituzione. Quanto poi all'attributo di rilevanza, basterebbe ricordare una norma che storicamente lo evoca proprio sul piano della offensività: il delitto di falsa testimonianza laddove, all'interno dei fatti apparentemente conformi al tipo, soltanto le false dichiarazioni che siano rilevanti perché davvero in grado di offendere il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia nel suo percorso di ricostruzione dei fatti per come effettivamente si grazie a tutto dell'attributo rilevante connesso a fatti materiali si pone nell'alveo storico del principio di offensività, nessun problema di costituzionalità si può porre perché questo attributo ha il pregio di ribadire la circostanza che non si puniscono fatti apparentemente conformi al tipo, ma in realtà non offensivi, che in questo contesto si possono presentare. È chiaro che sarà poi l'interpretazione dell'autorità giudiziaria a risolvere il problema. Ma non vi si possono calare quelle semplici valutazioni, estimazioni, quei falsi per errore che non sono in grado di determinare alcuna offesa del bene giuridico, vorrei dire quei falsi irrilevanti, per dimostrare con l'utilizzazione di un aggettivo contrario a «rilevante» proprio la portata dimostrativa dell'offesa implicata dall'utilizzazione dell'aggettivo «rilevante». Insomma, «rilevante» non è un qualsivoglia fatto, un fatto apparentemente conforme al tipo, ma non offensivo. «Rilevante» è proprio ciò che l'opposizione reclama debba essere un fatto di false comunicazioni sociali, un fatto effettivamente e concretamente in grado, in maniera rilevante, di ingannare i destinatari delle false comunicazioni sociali e che quindi, pur nel contesto di un reato costruito come reato di pericolo, si pone come reato di pericolo concreto.

pur promulgata prima e pubblicata poi, quindi dotata di esecutorietà, ma non ancora entrata in vigore, perché gli emendamenti non toccano questo aspetto, toccato però dalla pronuncia di questa Assemblea, che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità, potremmo dire quella che era stata posta con la seconda questione pregiudiziale di costituzionalità. Intervengo invece su una questione che ieri ha costituito oggetto di alcune considerazioni negative paradossalmente - e mi sia consentito questo avverbio - poste da una opposizione che invocava una struttura più garantista del testo della norma, entrando in conflitto, questa parte della opposizione, con le stesse premesse dalle quali si partiva. come ho detto in Commissione, ma mi permetto molto umilmente di riferirlo anche all'Assemblea, svolge una ulteriore, importante funzione selettiva della punibilità, quale prospettiva alla quale l'avverbio potrebbe tendere, potrebbe risultare funzionale ad escludere la forma più tenue di dolo, ossia il cosiddetto dolo eventuale, evocando non una consapevolezza del rischio di un evento, ma dicendo che il soggetto deve essere perfettamente consapevole del fatto, quindi non di un rischio di evento, ma della sua condotta. L'avverbio funziona, in tal modo, nella direzione della riduzione del campo di applicazione della norma e non certo nella contraria direzione della dilatazione della sua applicazione. Peraltro, com'è noto, il dolo ha un versante sostanziale, ma anche un versante processuale, come tutte le componenti delle fattispecie astratte di reato. L'avverbio implica ed in un certo senso richiede una dimostrazione ampia della consapevolezza del fatto e quindi funziona anche da elemento probatorio, da indice di una certa necessità di dimostrazione della consapevolezza del fatto. Quindi, in un certo senso marca ancora di più quello che è un generalizzato, certamente esistente, obbligo di motivazione del giudice su tutte le componenti della fattispecie, comprese le componenti di natura soggettiva.

Nel corso della discussione, è stato frequentemente affermato che l'efficacia di prevenzione generale connessa agli incrementi sanzionatori è dubbia, e quindi resterebbe privo di ogni effetto e di ogni funzionalità un incremento sanzionatorio che non darebbe, dal punto di vista della dissuasione, alcun Concordo su un aspetto: noi non disponiamo scientificamente di dati dimostrativi di una correlazione e della misura, tra l'altro, di questa correlazione tra gli incrementi delle sanzioni e l'eventuale dissuasione dal commettere reati di questo tipo.

ma trova una sua giustificazione ancora più storica e risalente sul versante retributivo. Intende dire il relatore che più crescono nella società l'intolleranza ed il rifiuto di determinati reati, maggiore è la giustificazione agli incrementi sanzionatori. Il legislatore allora, nella gerarchia del rilevante, nel selezionare i fatti deve anche risultare sensibile rispetto al crescente rifiuto sociale che si manifesta nei confronti di determinati fatti di reato. Più cresce la reazione sociale nei confronti di determinati reati, maggiormente si giustifica l'incremento sanzionatorio; ripeto, non sul versante della prevenzione generale, ma sul versante della retribuzione, di ciò che giustifica, secondo un detto che risale al 1500 e ad Ugo Grozio, l'incremento del trattamento sanzionatorio. C'è di più.

si scopre la connessione di questi reati con beni come l'economia nazionale, l'immagine internazionale del nostro Paese, della nostra Nazione, grazie a tutto se il reato è plurioffensivo, se si scopre che esso offende ulteriori beni giuridici, l'incremento sanzionatorio è giustificato anche su questo secondo versante.

signori senatori, vorrei innanzitutto ringraziare i componenti della Commissione giustizia che hanno contribuito ad elaborare, comunque a discutere e a modificare, e - a mio avviso - a migliorare il testo normativo oggi al nostro esame per l'approvazione. Voglio ringraziare poi tutti i senatori intervenuti nel dibattito perché credo abbiano dato un contributo alla riflessione e alla deliberazione che verrà di qui a breve. Credo che questa discussione, così come il lavoro svolto in Commissione, faccia giustizia di una polemica che è stata condotta contro questo ramo del Parlamento accusato di neghittosità o di volontà di non affrontare un tema rilevante come quello della corruzione. Penso sia una campagna sbagliata, ingiusta, sbagliata, ingiusta, che prescinde da un dato e cioè che un testo normativo diventa legge quando si compongono le condizioni perché quel testo sia sostenuto dai numeri necessari per diventare legge. E ciò avviene quando si risolvono delle contraddizioni politiche

di avere ricomposto posizioni diverse, a partire dalla propria posizione che era quella deliberata nel Consiglio dei ministri del 29 agosto. È stato fatto un rilievo, e cioè che poiché - come credo sia noto - sono convinto dell'esigenza di superare il bicameralismo sarebbe una contraddizione il fatto di aver sostenuto che alcuni provvedimenti approvati dalla Camera dei deputati possano essere migliorati nel passaggio parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento. È, a mio avviso, un rilievo paradossale perché noi legiferiamo con l'impianto costituzionale del quale disponiamo e non con un altro. Anzi, mi pare che chi muove questo rilievo mi rimproveri di non avere già abolito io, di fatto, il bicameralismo credo che questo sia francamente un rimprovero ingiusto. Io sono consapevole del fatto che aumentare le pene non basta e talvolta è inutile. E sono anche consapevole del fatto che talvolta la via più semplice per esorcizzare fenomeni profondi di grave allarme sociale sociale sia quella dell'inasprimento delle pene o quella dell'estensione dell'area del diritto penale. È un rischio che si corre sempre, quando si affrontano temi che sono posti dalla cronaca, e che diventa ancora più grave nei periodi di crisi sociale, come quello che stiamo attraversando. È un rischio che è anche indotto dal fatto che la possibilità di cimentarsi con alcuni temi dà un grande risalto mediatico. Ma questo rischio, che abbiamo corso, ha prodotto un testo che va in questa direzione oppure tale rischio è stato scongiurato? Ci siamo limitati ad inasprire le pene o abbiamo fatto qualcosa di diverso? Io credo che questo rischio, che abbiamo corso, sia stato scongiurato, perché non ci siamo limitati ad inasprire le pene. Eppure, anche sul tema delle pene una riflessione va fatta, riprendendo le argomentazioni del relatore. Nel corso di questo ventennio sono state enormemente inasprite le pene per i reati contro il patrimonio.

Significa che non cresceva la riprovazione sociale nei confronti di questi reati? Io penso di no. Significa, a mio avviso, che il legislatore aveva compiuto, in qualche modo, una scelta di campo, che noi abbiamo voluto mettere in discussione.

meno gravi (o considerati tradizionalmente meno gravi) e quello più grave della corruzione in atti giudiziari è una forbice relativamente contenuta. Noi siamo intervenuti per registrare un dato: cosa c'è di più grave, in un momento come questo, in un momento come questo, del comportamento di chi, svolgendo funzioni pubbliche, tradisce la comunità per realizzare un arricchimento improprio? E abbiamo dato una risposta a tale quesito. Certo, il diritto penale deve essere caratterizzato da efficacia e da congruità; ha anche una valenza simbolica e deve svolgere anche la funzione di registrare la riprovazione sociale che, in una determinata fase storica, si determina nei confronti di un comportamento.

con una volontà, che però è quella - e qui arrivo ad affrontare il resto del rilievo che è stato fatto di dare strumenti più efficaci e più congrui nel contrasto alla criminalità economica e mafiosa e nella lotta alla corruzione. Quando abbiamo iniziato questo percorso, le organizzazioni internazionali ci segnalavano dei vuoti. Ha ragione la presidente Finocchiaro: io sono assolutamente convinto che sia sbagliato rappresentare il nostro come un Paese privo di strumenti per la lotta alla corruzione. La semplice riprova è il fatto che molte inchieste dimostrano che esistono strumenti efficaci che consentono di intervenire in fenomeni di carattere corruttivo, le organizzazioni internazionali - non una parte o tutta la magistratura, non una parte dell'opinione pubblica o una parte della stampa - ci segnalavano che nel nostro Paese esistevano due gravi lacune: la prima era l'assenza dello strumento dell'autoriciclaggio; la seconda era un sostanziale svuotamento del reato di falso in bilancio. Intervenendo, prima nel testo sul rientro dei capitali e oggi con questo provvedimento, colmiamo queste due lacune. Con il reato di autoriciclaggio introduciamo uno strumento che consente di evitare le infiltrazioni nell'economia legale dell'economia criminale; che consente di evitare anche le conseguenze di una legislazione pregressa, che faceva sì che alcuni illeciti sostanzialmente provocassero un arricchimento contro il quale era impossibile esercitare la facoltà punitiva dello Stato. Oggi con l'autoriciclaggio alcune condotte che si prescrivono per i reati presupposto sono però perseguibili attraverso questo tipo di strumento. Con il falso in bilancio non tuteliamo semplicemente la società da condotte che sono il presupposto all'attività di carattere corruttivo; tuteliamo il mercato e l'economia nazionale e introduciamo un elemento di trasparenza anche per gli investimenti esteri. Ci siamo limitati sul 416-*bis* a inasprire le pene? No. Abbiamo ricostruito una figura che tiene conto dell'evoluzione del fenomeno della criminalità organizzata. Oggi la criminalità organizzata non è più soltanto quella che è cresciuta e si è sviluppata nel nostro Paese. Spesso è fatta di reti internazionali, dell'incrocio di mafie che vengono anche da altri Continenti, e oggi il 416-*bis*, così come è stato ridefinito, tiene conto di questa evoluzione storica. Abbiamo introdotto strumenti che incentivano la collaborazione che incentivano la collaborazione di chi è stato protagonista del patto corruttivo. Il presidente Palma si chiede chi mai mai romperà questo patto in cambio di una scelta del legislatore che consente di attenuare la pena; sostanzialmente manifesta un dubbio - così ho capito, altrimenti mi scuso altrimenti mi scuso - rispetto alla possibile efficacia di uno strumento come questo. Devo dire che, in questo caso, non soltanto una legislazione premiale in questa direzione ci è stata sollecitata da molti soggetti sovranazionali, ma in fondo l'esperienza della lotta alla criminalità organizzata ci dice che strumenti che incentivano la rottura del patto, che è il presupposto dell'attività di carattere criminale, la condizione anche per sconfiggere reti che ormai non sono più il frutto semplicemente di un rapporto sinallagmatico tra corrotto e corruttore, ma sono assai più complesse e fanno sì che oggi si possa dire che tra mafia e corruzione vi è una sostanziale sovrapposizione per le modalità attraverso cui il fenomeno si manifesta. Ho ascoltato con interesse, e senza alcuno spirito di chiusura, una sottolineatura che il presidente Palma ha fatto, cioè quella dell'esigenza di una presa d'atto del fatto che ormai i fenomeni corruttivi si sviluppano a livelli diversi, in campi diversi e anche con fenomenologie diverse. Devo dire che non ho colto una parallela iniziativa e una proposta che lavorasse sulla distinzione - se ho bene capito - tra grande corruzione e corruzione ordinaria,

all'evoluzione dei fenomeni di carattere criminale, debba essere fatto, realizzato e colto. Da questo punto di vista, trovo incongruo il continuo richiamo a termini come ribasso e rialzo, compromessi al ribasso e compromessi al rialzo. Lo dico perché credo che tutte le norme siano in fondo un compromesso tra esigenze di carattere diverso: tutte le norme tengono conto di un'esigenza di carattere punitivo, ma anche del fatto che lo Stato non può avere una funzione tanto invasiva da sconfinare nello Stato di polizia; tutte le norme devono tenere conto del fatto che da un lato si deve garantire la trasparenza del mercato, ma d'altro canto non si può neanche costruire degli strumenti che alla fine, nell'esercizio dei controlli, impediscono l'attività di mercato. Tutte le norme, nel loro intimo, sono il punto d'incontro di esigenze di carattere diverso, che talvolta sono manifestate da settori politici diversi, talvolta sono contenuti nell'animo stesso di chi propone la norma. Da questo punto di vista, il rialzo e il ribasso non può essere una valutazione di quanto alta è la pena, ma deve essere di quanto congruo e funzionale è l'insieme del sistema che si riesce a produrre: io credo che siamo riusciti a migliorare e a rendere più congruo e più funzionale il sistema di repressione di cui disponiamo. Come ho detto in più interviste, ma non amo autocitarmi, sono assolutamente convinto che la repressione sia soltanto una parte della lotta alla corruzione; forse una parte neanche determinante e lo vorrei dire nonostante il fatto che arrivare a un passaggio fondamentale consiglierebbe una certa enfasi propagandistica. Ma il fatto che si debba fare una prevenzione non è un buon motivo per non fare una seria analisi di ciò che non funziona nel sistema di repressione ed io credo che questo abbiamo fatto nel momento in cui si è compiuto questo tipo di elaborazione.

quanto di averlo attivato, perché in assenza degli strumenti previsti, in particolar modo dell'Agenzia,

il punto di riferimento di questo percorso di prevenzione. Abbiamo risolto tutto? No credo di no, perché, come tutti gli strumenti di prevenzione, è necessario evitare il rischio del «copia e incolla». Mi spiego. Noi siamo intervenuti in altri ambiti: penso a quello della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Spesso le pubbliche amministrazioni e le aziende hanno interpretato quest'onere semplicemente come un onere di carattere burocratico, risolto appunto attraverso lo strumento dei copia e incolla che venivano riprodotti in modo Dobbiamo invece fare in modo che i piani di prevenzione tengano effettivamente conto della specificità di quella realtà; tengano conto delle*performance* della pubblica amministrazione. Ma questo non lo garantirà alcuna legge: questo lo realizzeranno soltanto le forze sociali, i cittadini, le forze politiche e chi è chiamato a svolgere i pubblici uffici in concreto. Nessuna legge potrà garantire che quel percorso di prevenzione sia efficace e vivo, valutazione *ex post* che consente di verificarlo, che è il frutto di una dialettica sociale, di una capacità di vigilare, di una capacità di stimolare l'evoluzione delle pubbliche amministrazioni. La semplificazione è un obiettivo che questo Governo persegue, però attenzione, non vorrei nemmeno che questo argomento porti a dire che, siccome le norme sono molte complicate, allora bisogna essere bisogna essere indulgenti con chi le aggira utilizzando degli strumenti di carattere corruttivo, l'argomento della semplificazione è stato il presupposto alle deroghe e agli interventi di carattere speciale che hanno prodotto i vari campionati mondiali di nuoto, le varie ricostruzioni, Semplificare è un conto, considerare le norme e i controlli come un fardello inutile è un altro. Purtroppo questo Paese ha conosciuto questa seconda strada, che non è quella della semplificazione, ma che è quella della costruzione di percorsi di carattere eccezionale che sono stati assolutamente il presupposto allo sviluppo e alla realizzazione di fenomeni di carattere corruttivo. Vorrei concludere sottolineando un aspetto. So che, essendo alta la rilevanza simbolica degli interventi nel campo penale (e in un campo come questo, ci sarà sempre chi dirà che non si è fatto abbastanza e ci sarà sempre chi dirà che il problema è un altro. Noi lo abbiamo registrato in questi giorni: via via che si procedeva all'elaborazione del testo, «fuori» c'era chi diceva che vi era anche qualcos'altro da Non mi illudo che questo dato sarà risolto e superato dal voto di quest'Assemblea e neppure dal testo finale che uscirà dal Parlamento. su questo fronte, se davvero lo si considera un'emergenza di carattere nazionale, lo sforzo per la ricerca dell'unità dovrebbe essere il presupposto fondamentale dell'azione di tutte le forze politiche. Questo Paese ha sconfitto i fenomeni più gravi, dalla crisi economica derivante dalle macerie della guerra, al terrorismo, all'aggressione mafiosa nei confronti dello Stato, nessuno, credo, possa smentire questa mia affermazione - realizzare un grado sufficiente di unità di tutte le forze politiche. Noi non sconfiggeremo la corruzione e non riusciremo a dare un segnale chiaro, anche dal punto di vista culturale,

se continuiamo con polemiche di carattere pretestuoso, se continua la logica del "più uno", se continua la logica di smarcarsi rispetto al singolo punto sul quale non si è d'accordo, trasmettiamo un messaggio implicito all'opinione pubblica: si dice che si tratta di un'emergenza di carattere nazionale, ma poi si preferisce - in fondo - provare a lucrare qualche voto piuttosto che affrontare tale emergenza di carattere nazionale. Credo che vi siano le condizioni - per come fin qui si è sviluppato il dibattito - per fare un significativo passo in avanti, per togliere anche molti alibi e, davvero, per far sì che il Parlamento ponga al centro della propria azione il controllo e il monitoraggio sull'attività di prevenzione e di semplificazione.

avremo dato una risposta credibile a tutti i rilievi che il contesto internazionale ha posto alla nostra legislazione e a tutti i limiti che ha segnalato. Si valuti da questo punto di vista il provvedimento che stiamo per votare: rispondiamo in modo congruo a tutti questi rilievi. So che non sempre si tratta delle tavole legge di Mosè. Talvolta le organizzazioni internazionali seguono anche criteri che possono essere discutibili e opinabili, ma un'economia globalizzata non può sottrarsi a quel metro di giudizio. Facendo questo passo, accettiamo quel metro, facciamo un passo avanti e risolviamo una serie di contraddizioni presenti nel nostro sistema.

Mi auguro fino in fondo che su questo terreno cessi la propaganda e si riesca a fare qualcosa che concretamente contrasti il fenomeno corruttivo.

la Presidenza avverte che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell' articolo 113, comma 4, del Regolamento, su numerosi emendamenti, nonché su alcuni articoli del testo del disegno di legge in esame. In particolare, la Presidenza ritiene di non poter ammettere tale richiesta con riguardo all'emendamento 9.307, che ha un contenuto meramente processuale, in quanto limita la procedibilità a querela dei soggetti offesi ai ai soli casi di cui al secondo comma dell'articolo 2621-*bis* del codice civile, che concerne l'attenuante del fatto di lieve entità. La richiesta risulta invece ammissibile con riguardo agli emendamenti 1.1, 1.302, 1.19, 1.22, 1.321, 1.323, 1.326, 1.328, 1.330, 1.331, 1.333, 1.335, 1.341, 1.342, 2.301, 2.303, 3.0.301, 4.300, 4.302, 4.305, 5.300, 8.316, 8.327, 9.316, 9.317, 9.318, 9.320, 10.311, 10.317, 10.320 e 10.321, che attengono alle materie di cui agli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione. Per le stesse ragioni risulta altresì ammissibile la richiesta di votazione a scrutinio segreto degli articoli 1, 2, 8, 9 e 10.

meccanismo premiale per chi opera una condotta di tipo collaborativo al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

e che è vero che chi collabora spesso ha commesso un reato, riteniamo di dover incentivare chi intende dare il proprio contributo affinché siano scoperti

particolari che fanno venir meno proprio la fiducia stessa nelle istituzioni non debba avere la possibilità ancora di contrattare con la pubblica amministrazione vista in sé la pericolosità della sua condotta.

vergognoso per chi opera all'interno dell'amministrazione. Noi siamo affinché la pubblica amministrazione debba sempre comportarsi con condotte assolutamente ineccepibili e riteniamo che chi opera dietro ad uno sportello, qualsiasi esso sia, debba improntare la propria condotta a particolari criteri di rigore.

del Consiglio Renzi. Sulla dichiarazione di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione da parte di chi si è reso colpevole, a fronte di una sentenza passata in giudicato, di reati gravi e gravissimi nei confronti della pubblica amministrazione c'è stato un dietrofront per la verità del tutto inaspettato, inatteso e ingiustificato da parte della maggioranza e Governo in Commissione giustizia. Aula potremmo solennemente richiamare l'attenzione della maggioranza rispetto a questo importante provvedimento, perché la situazione della corruzione nel nostro Paese è emergenziale ed è necessario intervenire con strumenti che siano

ma anche Astorre, Capacchione, Cirinnà, Cuomo, D'Adda, Fedeli, Gatti, Rita Ghedini, Guerrieri, Mineo, Moscardelli, Parente, Puglisi, Puppato, Saggese, Scalia, Sollo, Zanda, Bubbico, Di Giorgi, Lucherini, Favero,

Concludo con una richiesta a Governo e maggioranza di modificare il loro parere.

i reati oggetto del disegno di legge con l'istituto della prescrizione. Alla luce dei noti fatti legislativi della Camera, onde evitare ogni tipo di confusione e sovrapposizione, preferiamo ritirarli in questa sede.

ha, per più aspetti, modificato in senso peggiorativo le pene principali ed accessorie previste per i reati contro la pubblica amministrazione. L'obiezione non dovrebbe sembrare secondaria, per due ordini di ragioni. Innanzitutto, le pene prevedute dalla legge sopra richiamata sono state recentissimamente ritenute congrue dalle medesime forze politiche che oggi dovrebbero decretarne un ulteriore inasprimento. Sfuggono, tuttavia, le ragioni giustificative di una simile scelta la quale, secondo corretti criteri di politica criminale, dovrebbe fondarsi sulla constatata e palese inadeguatezza del precedente inasprimento sanzionatorio. Sul punto, a parte l'ovvio a parte l'ovvio rilievo secondo il quale nessuno riesce a comprendere per quale motivo dovrebbe essere incongrua la pena ad anni "x" di reclusione, laddove sarebbe congrua la diversa pena ad anni "x più uno", non si comprende quale evidenza politica criminale possa aver segnalato l'erroneità delle scelte appena compiute dal Parlamento, dato che se ne registra ancora un'attuazione talmente ricca e dimostrativa della sua eventuale inefficacia da giustificare una modificazione così frettolosa. Né, peraltro, andrebbe trascurato il principio costituzionale che impone un necessario rapporto di proporzione tra gravità del fatto ed entità della relativa sanzione».

quando ha affermato che a suo avviso l'aumento delle pene non sempre costituisce un'adeguata deterrenza al reato di corruzione e che anzi talvolta è anche inutile,

Aula, lavoriamo per contrastare la corruzione. Il problema è che ciascuno di noi può percorrere strade differenti:

grazie a tutto certamente di emendamenti che vanno nella direzione di favorire o di sopportare e giustificare

alzano, ma di effetti sostanziali di contrasto al fenomeno della corruzione. Detto questo, desidero invitare il Ministro e il Governo a fare una riflessione. Se è vero, signor Ministro, che ella ritiene che l'aumento della pena

e prenda in considerazione l'eventualità di percorrere anche la strada della prevenzione, che peraltro non è in contrasto anche con la vostra posizione di inasprimento della pena.

1.309. Si tratta della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale ovvero di un'arte. In concreto si chiede un aumento del minimo e del massimo, da quindici giorni a tre mesi e da due anni a tre anni.

La riformulazione dovrebbe sostituire le parole «fino a due terzi»

Signor Presidente, l'emendamento 1.308 ha l'obiettivo di segnalare una problematica importante, tra l'altro ripresa anche dal ministro Orlando, che è quella del rapporto fiduciario tra i funzionari della pubblica amministrazione e i cittadini.

al fenomeno corruttivo non può rappresentare un punto di riferimento futuro nella pubblica amministrazione. L'emendamento tendeva a segnalare la necessità di un maggiore severità rispetto ai comportamenti dei pubblici funzionari. Prendo tuttavia atto delle considerazioni del Ministro e lo ritiro.

quando dice che le forze politiche numericamente più rilevanti in quest'Aula surrettiziamente ritirano gli emendamenti un minuto prima del voto. A parte che questa considerazione può essere rivolta solo ed esclusivamente al Partito Democratico, mi permetto di dire al senatore Cappelletti, sperando che l'entusiasmo non lo faccia distrarre, che ha fatto propri gli emendamenti del senatore Casson 1.312 e 1.313 che sono similari agli emendamenti 1.310 e 1.311 del senatore Buccarella, cioè del Movimento 5 Stelle, poco fa ritirati esattamente dal presentatore.

per poter verificare che quello che ha sorprendentemente sostenuto il presidente Palma non corrisponde a verità. Infatti, il contenuto degli emendamenti da lui citati è completamente diverso, attenendo la portata degli emendamenti fatti propri dal Movimento 5 Stelle all'istituto della prescrizione

che l'altro ramo del Parlamento, la Camera, avesse approvato un disegno di legge che interviene proprio sulla prescrizione. La scelta del Governo è stata quella di una linea rigorosa

Signor Presidente, vorrei che tutti prestassero attenzione a questo emendamento. Ho solo proposto la diminuzione della pena minima, mantenendo la pena massima che era stata proposta dal Governo. Non devo insegnare al presidente Grasso che questo rientra nelle logiche della tecnica normativa in materia penale, che lascia al giudice la possibilità di valutare fatti minimi. Stiamo trasformando, con queste norme, la nostra giustizia in una giustizia della misura cautelare, come ha detto il professor Flick qualche giorno fa: una giustizia della misura cautelare e non di accertamento della responsabilità, per affermare quali sono le vere responsabilità e qual è la pena graduata a seconda della gravità del fatto. Se noi partiamo da sei anni, in un sistema penale dove questa pena non è prevista, vi rendete conto che una pena minima di sei anni rende impossibile qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice. E veramente quella giustizia della misura cautelare e non più della responsabilità penale l'avremo già realizzata.

La finzione che le pene del codice penale siano quelle edittali o quelle massime è intollerabile soprattutto da parte di soggetti che hanno buona dimestichezza con le aule di un tribunale e, quindi, sanno bene quanta influenza ha il minimo della pena, che è quella che si discute realmente nelle aule, e che i minimi edittali non sono mai quelli che vengono erogati, grazie a tutto quel complesso di norme processuali e di percorsi alternativi imbastiti negli ultimi anni.

il senatore Caliendo voterà a favore dell'emendamento 1.321, mentre io personalmente mi asterrò, perché non intendo in alcun modo partecipare ad una Senato-vendita che è rappresentata da questo provvedimento. Il punto in discussione è molto semplice: il Ministro, nella sua replica, ha riconosciuto che probabilmente l'intervento in tema di corruzione poteva essere diverso. cioè, immaginare una modifica legislativa riguardante la corruzione nei grandi appalti, nelle grandi opere, ovvero quelle opere in cui alberga il cosiddetto sistema corruttivo. E sotto questo profilo aveva e ha un senso la legislazione premiale, pur introdotta in questo testo. Per converso, si poteva lasciare inalterata o - se si vuole - inasprire ulteriormente le pene per la corruzione e gli altri reati della pubblica amministrazione riguardanti opere diverse da quelle fondamentali per la modernizzazione del Paese. Questo non si è voluto fare. Si è fatto di tutta l'erba un fascio. Si è immaginato che questi reati fossero solo contro la pubblica amministrazione e non anche contro l'economia nazionale e, con scarsa fiducia

Sicché, al di là della posizione espressa poc'anzi, secondo il suo solito stile, dal senatore Giarrusso, si è immaginato che il reato di corruzione avesse un minimo di sei anni. la corruzione non è solo quella del MOSE o dell'Expo, dei grandi appalti o di Mafia Capitale. È anche la corruzione - se mi passate il termine - straccionesca,

per superare il passaggio della Corte costituzionale, deve avere una sua razionalità, e questa si fonda sulla proporzionalità tra la pena, in concreto e in astratto, e il fatto realmente commesso, mi chiedo e vi chiedo: scusate, ma voi ritenete razionale e proporzionale che un giudice, come è sempre accaduto, nel passaggio tra i minimi e i massimi della pena, condannare un soggetto che, per ipotesi, ha commesso un reato di corruzione per 1.000 euro, ad una pena - sbaglia il senatore Giarrusso - che, ove mai gli si dovesse riconoscere un'attenuante, ove mai si dovesse percorrere un rito speciale, sarebbe certamente superiore ai due anni e sei mesi e, quindi, sicuramente foriera del carcere? Il riportare - questo dice l'emendamento - il minimo della pena da sei a quattro anni, lasciando completamente inalterato il massimo dei dieci anni, significa soltanto dire al giudice che, di fronte ad un episodio grave di corruzione, ma rispetto a tutti gli altri episodi di corruzione sicuramente marginale, di irrogare una pena più adeguata al fatto concreto commesso. Con l'emendamento in esame non vogliamo impedire una furiosa reprimenda di chi commette il reato di corruzione. Vogliamo semplicemente dare al giudice la possibilità di adeguare la pena che andrà a irrogare in concreto rispetto al fatto concretamente posto in essere dal soggetto.

Stiamo parlando del reato di corruzione, che è il cuore delle varie fattispecie che intendono intervenire e colpire i vari aspetti della corruzione. Colleghi, stiamo parlando della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio quindi, di un aspetto delicato ed importante della lotta alla corruzione. Abbiamo detto in Aula - e tutti siamo d'accordo - che non basta aumentare le pene, ma contrapporre l'aumento delle pene alla prevenzione è un errore, e un Paese avanzato, un Paese maturo, non lo commette. Quindi, bene ha fatto il Ministro nella replica a ribadire la necessità di una visione che integra la prevenzione con la repressione. Siamo pure tutti d'accordo che c'è bisogno - ed è stato detto in diversi interventi - di aumentare il tasso di intervento, attraverso altre procedure e vie, nella lotta alla corruzione. Abbiamo parlato di piano integrato sugli appalti - altroché - e di interventi sulla pubblica amministrazione, e questa è la linea che il Governo ha scelto e che il Parlamento deve seguire.

l'attuale legislazione prevede da quattro a otto anni. Quindi, si tratta di minimi aumenti di pena proporzionati, in grado di rispondere meglio, per l'aspetto specifico e limitato della repressione, a quello che ci è stato sottolineato. E il Presidente sa - e lo ribadisco - che con le attenuanti generiche e i riti speciali, il pericolo che paventava quando si tratta di fatti di poco conto può essere facilmente affrontato da parte del giudice e risolto brillantemente. Signor Presidente, io invece, a differenza del senatore Palma, voterò a favore di questo emendamento, anche se condivido *in toto* l'intervento svolto dal Presidente della Commissione. Lo condivido a tal punto che mi avrebbe posto dei problemi se il senatore Lumia non fosse grazie a tutto

Ma sapete capire quello che leggete o quello che dite? Sapete capire che, quando si parla di prevenzione, non si interviene tanto per buttare La prevenzione si fa negli atti, nei fatti. Cosa fa questo Governo per la prevenzione? Abbiamo fatto emendamenti per togliere la politica dalle ASL, dal coperchio che c'è sulla nomina dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi, dei primari, e avete detto di no. Avete detto, voi del Partito Democratico, con Lumia in testa, no all'emendamento del senatore Palma, prima, e mio e di Ciro

la pena minima, per far sì che 50 euro non siano paragonabili a 5 milioni. È un reato, lo condanniamo, ma diamo anche la possibilità di differenziare la pena da comminare in base alla gravità del fatto.

questo che vogliamo dire, né più e né meno. Ed è per questa ragione che convintamente voterò a favore di questo emendamento garantista, perché è questo che volevano i Padri costituzionali.

Presidente, ritiro la firma da questo emendamento e dichiaro di votare in dissenso. Ma lei mi deve consentire di precisare al senatore Lumia che non è affatto vero che non vi è differenza sul piano delle conseguenze. Il senatore Palma è stato molto chiaro nel precisare che la riduzione della pena per un reato contrario ai doveri d'ufficio, che può comportare un vantaggio o comunque un prezzo della corruzione di 500 o di 1.000 euro,

mi sarei dimesso dalla magistratura se fosse passata una norma come quella che abbiamo appena votato sulla corruzione.

posizione. Signor Ministro, con grande rispetto vorrei dirle che, avendo giurato fedeltà alla Costituzione, non avrei mai potuto applicare norme di questo tipo, perché ciò avrebbe significato, per forza di cose, mettere in galera persone che poi sarebbero state assolte. Questo è assurdo! So benissimo che ci sono stati magistrati che hanno accettato di restare tali pur dovendo applicare le leggi fasciste. Noi non possiamo arrivare a questa abnormità, alla aberrazione

e prima di me, ha fatto alcune affermazioni quando era Presidente della Camera proprio su questa materia.

per fatti minimali, ancorché gravi, e solamente per accuse ancora infondate e non controllate, facciamo arrestare anche degli innocenti.

Lei ricorderà i rilievi in sede europea al nostro reato di concussione, che impediva nell'applicazione dei Paesi europei di tener conto della responsabilità del concusso. E per questa ragione si arrivò ad una nuova formulazione. Il ministro Orlando ricorderà che, in una serie di incontri che ebbi come Sottosegretario con l'OCSE, dovetti garantire che questo Parlamento modificava la legge sulla concussione. Fu modificata e il Ministro ricorderà che uno dei migliori esperti di diritto penale del nostro Paese, la professoressa Severino, spiegò e diede conto delle ragioni per cui gli aumenti di pena, che propose e che furono attuati, dovevano rispondere ad un principio di equilibrio del sistema sanzionatorio. Ora, senza alcuna rilevata deficienza di funzionalità sotto il profilo della misura della pena, si passa da tre a sei anni nel minimo. Voi vi rendete conto delle persone assolte dopo un processo? Che dovremmo fare? Pensate di fare il magistrato per un giorno, per un'ora, ritrovate con una pena di sei anni nel minimo. Cosa fate durante le indagini? Arrestate o meno la persona? E poi avete il coraggio di assolverla, dopo avergli fatto scontare un anno di carcere,

Abbiamo previsto appositamente un reato di induzione, che può consistere anche in fatti minimi. Come si fa a dire che sei anni devono essere per forza erogati come minimo?

sull'aumento delle pene, che è un fatto vergognoso. Si arriva a prescrizioni che non possono essere tollerabili in base alla nostra Costituzione. Una prescrizione che dura 20 o 30 anni

di cui dobbiamo avere rispetto, e non per nostra scelta, ma in base all'articolo 2 della Costituzione, che proclama i diritti della persona. E voi volete mettere in galera o esporre al

Ministro, anche non condividendo l'aumento del massimo, ho chiesto solo la riduzione del minimo lasciando a lei, per quell'adeguamento cui ha fatto riferimento in relazione alla prescrizione, le scelte. Io non ho inciso sull'aumento della pena, ma lei salvi i principi del diritto penale, salvando il minimo.

tutto quanto detto dal senatore Caliendo. Ciò nonostante, invito a votare contro l'emendamento del senatore Caliendo, e ne spiego le ragioni. Tutto il problema che riguarda questa legge nasce da quell'emendamento del Governo che porta la pena della corruzione da sei a dieci anni. In ragione di questo, vi è stata la necessità di adeguare l'attuale sistema sanzionatorio sulla base di quell'emendamento del Governo. E non è un caso - ad esempio - che la corruzione impropria (cioè quella per atto del proprio ufficio) sia passata nel massimo a sei anni, anche se devo riconoscere che ciò era chiaramente piegato alla necessità di consentire delle intercettazioni telefoniche. Ma nella lettera *g)* vi è l'esempio lampante dello sconquasso che voi state combinando. Il professor D'Ascola, che ben conosce la materia, per cercare di razionalizzare il sistema sanzionatorio portare il minimo della pena della concussione per induzione allo stesso livello della corruzione propria e aumentare il massimo della pena della concussione per induzione a un tetto superiore a quello previsto dall'emendamento governativo, sicché - unico caso nel nostro codice penale - quando voterete questo emendamento, ci troveremo di fronte ad una pena

perché su questo emendamento il ragionamento della Corte costituzionale sarà evidentemente *tranchant*, visto che non è possibile immaginare che nel nostro codice vi sia un reato più grave, come la concussione per induzione, che abbia lo stesso minimo di pena della corruzione - ovvero sei anni - e abbia come differenziazione solo sei mesi in più nel massimo.

perché rientra sicuramente nella discrezionalità del legislatore conferire maggiore gravità ad un reato rispetto ad un altro

di quello di corruzione - e immaginare che la concussione per induzione sia un reato meno grave rispetto alla corruzione e, conseguentemente, ove mai si dovesse accogliere l'emendamento Caliendo, conferire una pena significativamente diversa dal reato di corruzione. So che queste sono tutte chiacchiere al vento e so perfettamente che la forza dei numeri numeri deporrà nel senso del varo di questo provvedimento. Le nostre, quando si sollevano, sono solo voci di testimonianza,

con un forsennato inasprimento sanzionatorio, se così si vuol fare, ma rispettando i criteri e i dettami propri del nostro ordinamento costituzionale e del nostro ordinamento di settore. Non diciamo nient'altro che questo. Siamo consapevoli del fatto che questa legge non avrà una grande vita, perché la maggioranza non ha inteso e non intende accogliere quei piccoli contributi di buonsenso, quei piccoli contributi giuridici, se volete, che stiamo cercando di portare dai banchi dell'opposizione.

dalle sue articolazioni referenti. Solo questa è stata la ragione di quell'ostruzionismo, che non a caso è cessato nel momento stesso in cui è stato depositato quell'emendamento. Non stiamo facendo ostruzionismo, non stiamo parlando su tutti gli emendamenti, ma solo su quei tre o quattro emendamenti che a nostro avviso - forse è sbagliato - denunciano un'assenza di misura nel sistema sanzionatorio, con riferimento ai fatti concreti che il giudice può trovarsi davanti e denunciano altresì una scarsa razionalità nella comparazione delle sanzioni, che assistono delle figure di fattispecie criminose tra di loro assolutamente diverse. Tutto qua. Vi stiamo chiedendo di andare avanti con le vostre idee, di votare i vostri provvedimenti, ma quanto meno di blindarli dalle inevitabili dalle inevitabili questioni di legittimità costituzionale che li aggrediranno e che porteranno questa legge, di qui a breve, ad essere seriamente aggredita e toccata dalla Corte costituzionale.

più lunga per continuare a torturare i nostri cittadini, a vessarli, a dire loro che sono schiavi perché c'è qualcuno che si impone e riesce a dominare la politica e qualsiasi amministrazione, scegliere chi indagare

Nell'Italia di Mussolini era in vigore il codice Rocco, molto ma molto più garantista di quelli che abbiamo adesso.

ai Padri costituenti chiedendo loro di perdonarvi per il male che state facendo ai loro sforzi e al sangue che hanno versato per liberare l'Italia e darci una democrazia che adesso viene calpestata. Padri costituenti, perdonate loro che non sanno il male che fanno!

mi permetto di intervenire sulla questione delle sanzioni, soprattutto con riferimento ai minimi edittali.

fondatezza di talune questioni che inevitabilmente sorgevano in conseguenza del fatto che il Governo aveva trasmesso un emendamento il quale incrementava la pena minima per il delitto di corruzione, corruzione propria, ossia per atto contrario ai doveri dell'ufficio. Tutti sappiamo che sia nel testo base del disegno nel testo unificato che io avevo preparato, la pena minima era di quattro anni e la pena massima era di dieci anni. Ciononostante, è chiaro che per la maggioranza l'orientamento di politica criminale del Governo non può certo essere considerato come un fatto irrilevante o trascurabile: è chiaro che, avendo il Governo dettato delle linee di politica criminale che si riflettevano in un incremento sanzionatorio, la maggioranza presente all'interno della Commissione giustizia non potesse manifestare atteggiamenti di indifferenza rispetto ad una rispettabile linea di politica criminale. C'è da osservare, e in ciò mi permetto di rispondere all'obiezione del senatore Palma, che non è vero che soltanto per questo caso sia prevista una pena, quella massima, che prevede il ricorso a frazioni di anni (anni dieci e mesi sei), perché non soltanto se si consulta la legislazione penale complementare, ma direi in particolare il codice civile in materia di reati societari, vi si scorgono pene le quali fanno uso di frazioni di anno, quindi di sei mesi di reclusione, per dettagliare meglio le pene. Mi permetto però di intervenire sulla questione di costituzionalità che è la più importante ed è quella che ha indotto il relatore ad intervenire nella direzione di un adeguamento che funzionasse come armonizzazione del sistema sanzionatorio per i delitti contro la pubblica amministrazione. Orbene, in questo noi abbiamo il supporto della Corte costituzionale, che in determinate vicende - ne cito una per tutte, quella relativa al delitto di oltraggio - ha affermato dei principi chiari: arbitro del trattamento sanzionatorio è il potere legislativo, questo è indiscutibile, perché si tratta di valutazioni di merito, di apprezzamenti che riguardano ovviamente la valutazione che il potere legislativo fa con riferimento alla gravità dei reati, in conseguenza della quale gravità dettaglia pene che siano proporzionate. Devo anche dire che le frontiere dal punto di vista della stima di una pena giusta, sono frontiere mobili: noi non possiamo pensare che valutazioni risalenti agli anni Trenta siano ancora oggi attuali, in conseguenza del mutamento della rilevanza penalistica, ma prima ancora sociale di condotte offensive di beni giuridici, che ovviamente assurgono a maggiore rilevanza in conseguenza di fenomeni sociali che non possono essere bloccati. senso, dobbiamo essere consapevoli della libertà del legislatore, il quale fa apprezzamenti di merito, ma che devono tener conto di quella gerarchia del rilevante che fa in modo che il legislatore debba esprimere valutazioni con carattere di attualità. Il limite di costituzionalità degli apprezzamenti che il legislatore svolge con riferimento alla pena che si ritiene giusta per coprire l'offensività ed il disvalore di quel determinato reato è una valutazione che può essere affetta da incostituzionalità se palesemente irragionevole: questo è il limite fissato dalla Corte costituzionale. Fatti allora salvi i casi di palese irragionevolezza, che il relatore si permette di ritenere da non riscontrarsi (poi è chiaro che ognuno può esprimere, e ci

superiore alla corruzione per una tradizione ancora difendibile, rilevante e attuale: si è sempre ritenuto che la famiglia - uso impropriamente questo termine, però oggi attuale dei delitti di concussione, ai quali indubbiamente l'indebita induzione appartiene sia pure nel livello meno grave del disvalore, meritasse comunque un segnale di maggiore gravità

Siamo dunque davanti ad un bivio e si è parlato a lungo, nei giorni scorsi, dell'attitudine di questo Parlamento, o meglio di questa maggioranza e dell'attuale Governo, a dare uno schiaffo ai magistrati e una carezza ai corrotti. Bene, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto fino a adesso. Abbiamo bocciato il DASPO per i corrotti e i corruttori. Abbiamo bocciato l'emendamento - non del Movimento 5 Stelle, ma presentato da esponenti della maggioranza - che imponeva il licenziamento del dipendente che commette reati contro la pubblica amministrazione con pena inferiore ai tre anni. Abbiamo bocciato una riforma della prescrizione che era stata da voi stessi proposta e che prevedeva la sospensione dal rinvio a giudizio oppure dal primo grado, sicuramente più avanzata ed efficace rispetto a quella che è stata votata recentemente nell'altra Aula del Parlamento. Sarebbe stata efficace per evitare nuovi casi Penati nel nostro Paese. inquirente uno strumento efficace d'indagine, cioè l'introduzione di un conflitto di interessi fra corrotto e corruttore. Abbiamo la possibilità di rompere dunque quel rapporto di correità, consentendo di far emergere reati cui, per la stragrande maggioranza, non si è mai a conoscenza. Non è solo una nostra proposta, non è solo una proposta del Movimento 5 Stelle, ma anche una vostra proposta (parlo del Partito Democratico), perché è contenuta nel disegno di legge Grasso sottoscritta da oltre 30 senatori del Partito Democratico, tra cui il capogruppo Luigi Zanda. Quindi abbiamo la possibilità di dare una risposta alla domanda iniziale: è vero quanto è stato dichiarato, cioè che la politica di questo Parlamento è di trattare con una carezza corrotti e corruttori e con uno schiaffo i giudici, intervenendo magari con una nuova norma più restrittiva sulle intercettazioni, visto e considerato che ci sono troppe inchieste che portano a galla eventi corruttivi nel nostro Paese? Spetta a voi dare una risposta; mi appello quindi a tutte le vostre coscienze.

Dicendo che i giudici prendono gli schiaffi e i corrotti le carezze, credo che siamo fuori tempo, fuori luogo e fuori spazio; e non aggiungo nient'altro.

Tutti i dati statistici dicono che siamo in preda ad un'epidemia che forse può portare alla morte il Paese. Ovviamente apro la cartella clinica di questa epidemia e prendo i dati, signor Presidente, che vengono dalla commissione costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica dall'allora ministro Patroni Griffi nell'ottobre grazie a tutto grazie a tutto

tutti i funzionari pubblici e tutti i pubblici dipendenti (4 milioni), compresi tutti i politici, siano corrotti, gli altri 5 milioni da dove vengono?

Senatore Barani, la invito ad un linguaggio consono a quest'Aula. I ceffoni li può dare fuori da qui, anche se sono metaforici,

Presidente, anche se l'ho accennato prima, vorrei che i presentatori mi ascoltassero.

e, anche dal punto di vista della normativa penale di riferimento, occorre tenere conto di quello che avviene in Europa e negli altri Paesi. L'OCSE per circa sei anni ha premuto sull'Italia perché fosse spacchettato il delitto di concussione che non prevedeva, come non prevede quando vi è la costrizione, la punibilità del concusso.

- e siamo riusciti, attraverso una delle poche norme che ha trovato l'accordo dell'intero Parlamento, ad individuare una punizione, non molto alta, diversa, rispetto a colui che commette il reato di induzione; reato di induzione; reato che è molto prossimo alla corruzione e non a quello della corruzione per costrizione. Per questa ragione sarebbe un errore madornale, anche dal punto di vista economico, nei rapporti e nelle influenze sull'economia nazionale, eliminare il comma

voglia dilatare - e ci mancherebbe altro - i tempi di discussione, ma perché questo è un punto qualificante. Tra l'altro, si riflette anche su taluni emendamenti presentati con riferimento all'articolo 2;

Il dibattito penalistico degli ultimi quindici anni in materia di reati di corruzione è stato occupato, per l'appunto, da quello che, con un brutto termine, si chiama lo spacchettamento della concussione, ossia organismi internazionali, tra i quali principalmente l'OCSE, rimproverano all'Italia, utilizzando il delitto di concussione, un'incompleta e inefficace tutela contro la corruzione. Si diceva Si diceva infatti: visto che avete la non punibilità del concusso (all'epoca era il concusso sia per costrizione sia per induzione), al corruttore risulterà agevole travestirsi da concusso per sottrarsi alla punibilità prevista per la corruzione. l'assetto della concussione, nel non prevedere alcuna punibilità per il concusso, indebolisce la corruzione. In questa direzione e in ubbidienza alle polemiche e ai richiami di questi organismi internazionali, nel 2012 si è ritenuto di separare la concussione per costrizione dalla concussione per induzione, creando per l'appunto l'articolo 319-*quater* che, nel suo secondo comma, prevede una pena, tra l'altro estremamente ragionevole, per colui il quale è stato indebitamente indotto (diciamo che è una sorta di concusso di serie B), per rimarcare la distinzione rispetto alla figura generalista di concussione per costrizione (che continua a mantenere la non punibilità del concusso per effetto di violenza o minaccia, quindi in una situazione di costrizione). A questo punto, l'emendamento proporrebbe un ritorno al passato. Non che al passato sia vietato tornare, per carità, ma se - ripeto - tutto il dibattito di quindici anni di diritto penale su questi temi è stato finalizzato a trovare una soluzione al problema, determinato dai richiami soprattutto dell'OCSE con riferimento a questa storica storica non punibilità del concusso e quindi dei riflessi di questa non punibilità sui delitti di corruzione, oggi il ritorno al passato non soltanto sarebbe privo di ogni giustificazione, ma si porrebbe in controtendenza, potremmo dire radicale, con quella che invece è una soluzione conforme a tutta una serie di indicazioni funzionali ad incrementare la punibilità dei delitti di corruzione Mi permetto di osservare che, tra l'altro, questo testo legislativo si compone anche di una norma che riguarda la collaborazione e gli effetti della collaborazione. La collaborazione ha una doppia faccia: è una circostanza attenuante per chi collabora,

utilizza l'avverbio «efficacemente» per sottolineare la circostanza che può godere dell'attenuante della collaborazione chi abbia dato comunque un contributo funzionale all'incremento dell'indagine, alla conservazione delle prove e del provento delle attività illecite, e comunque dell'evoluzione delle attività del pubblico ministero. ciò che si perde sul versante di quell'incremento alle indagini che poteva scaturire dalla non punibilità del concusso (che rimane non punibile perché qui parliamo della non punibilità dell'indebitamente indotto), lo si guadagna per effetto di una nuova circostanza aggravante, che però è funzionale all'incremento del patrimonio conoscitivo del pubblico ministero e delle indagini, della conservazione del materiale probatorio e anche della conservazione del profitto. È questa la ragione che, non soltanto con riferimento a questo emendamento ma anche a quelli che, con riferimento all'articolo 2, lambiscono comunque il problema della punibilità dell'indebitamente indotto, ha portato il relatore, ma anche il Governo, ad esprimere parere contrario.

un ragionamento su questo importante provvedimento, che - come dice il senatore Barani da medico - parte dalla diagnosi. Vorrei rassicurare i colleghi che i 60 miliardi di euro all'anno di corruzione da cui sarebbe afflitto il nostro Paese - che purtroppo ci hanno distrutto in tutto il mondo sul piano della reputazione - non esistono da nessuna parte. La Corte dei conti non ha mai detto una cosa talmente sproporzionata e fuori dalla realtà. Stiamo parlando, come il Governo dovette rispondermi in Commissione e in Aula due anni fa, della cosiddetta corruzione percepita e di un sondaggio di opinione che il Governo Monti commissionò interrogando i cittadini e chiedendo il loro parere su quale ritenessero fosse la corruzione del nostro Paese; è l'unico dato esistente. Infatti, se fossero davvero 60 miliardi di euro all'anno, sarebbero 600 miliardi di euro in dieci anni. Ricordo ai colleghi che, per fortuna, anche sulla base della normativa vigente, la magistratura ha scardinato

con l'Expo di Milano ed è intervenuta a Roma. Ma, facendo il conto di tutto quello che potenzialmente è stato - cose gravissime - versato in dieci anni in termini di corruzione, siamo a circa 100 milioni

i finanzieri o i carabinieri che si fanno corrompere e ci sono quelli perbene. Prego, allora, i colleghi di non fare dell'autolesionismo, perché paragonarci perché paragonarci ai Paesi del Terzo mondo e ai più corrotti dell'Africa mette questa realtà totalmente in contrasto con quella che è l'effettività di un fenomeno pur grave, che giustamente combattiamo.

dal nostro autolesionismo nazionale, dal nostro parlarci addosso, dal nostro pessimismo e che raffigurano una realtà che, fortunatamente, è curabile, se si interviene con decisione

che misure di questo tipo furono proposte dal compianto Michele Coiro e dal sottoscritto all'epoca del terrorismo in sede di Consiglio superiore della magistratura.

l'individuazione del pentitismo in questa materia perché credo ancora, forse sbagliando, in uno Stato che, attraverso la norma,

i valori in cui credo: un legislatore deve emanare norme che siano indicative di quale sia il modello di cittadino che rispetta la legalità,

utilità diverse come incarichi professionali o chi va a braccetto con qualche esponente della mafia si fa fotografare con queste persone. Questa, signor Presidente, è la realtà. E allora dare soltanto a queste persone la possibilità di avere una riduzione della pena era una cosa che mi dava fastidio. Io avrei preferito norme chiare, equilibrate, che dessero un'indicazione seria di lotta alla corruzione ma, allo stesso tempo, dessero un'indicazione ai cittadini di cosa sia la legalità e di come bisogna comportarsi nel vivere civile.

fai pure quello che devi fare, poi ti penti e dai un contributo individuando qualcun altro dei responsabili. È una cosa un po' vergognosa,

giudiziario, ci riporta dei numeri che sono solo percepiti. Quando dice che la corruzione è 60 o 100 miliardi l'anno, dice delle cose percepite e non reali? È di una gravità inaudita.

bisogna intervenire immediatamente perché un organo dello Stato non può fare questo contro il suo Paese.

per certa sinistra, per il terrorista Cesare Battisti, non è valido. Deve essere libero in Brasile. Invece, due ragazzi che hanno fatto il loro dover, i marò che sono in India, sono in carcere per terrorismo.

*in dubio pro reo*. Visto che siamo stati la Patria della cultura con questo grande popolo duemila anni fa, cerchiamo di portarla avanti in questo Parlamento più garantista e meno giustizialista.

Ci siamo interrogati in questi anni, nella lotta alla corruzione, su come spezzare il vincolo che si viene a creare tra corrotto e corruttore. Nel nostro Paese, unico caso tra i Paesi avanzati, abbiamo storicamente un'altra fattispecie, quella della concussione. anche lì ci si è chiesti come spezzare questo vincolo. E questo vincolo era spezzato dalla possibilità del concusso di dare dare un contributo, di scaricare la responsabilità penale e di fare in modo che, attraverso una delegata responsabilità, potesse aggirare i rigori della legge. È vero. Su questa fattispecie a livello internazionale ci sono stati molti rimproveri al nostro Paese. Addirittura siamo eliminare il reato di concussione, a trasferire tutto sulla corruzione e, attraverso la ridefinizione del reato della concussione e delle aggravanti, a ricomprendere e colpire tutti i soggetti protagonisti della corruzione.

che, storicamente, aveva dato in fase d'indagine alcuni risultati: al di là della valutazione che su questi risultati si potesse formulare.

Avevamo un'altra via, che valuteremo dopo: quella dell'agente sotto copertura, previsto dal nostro codice. Tale figura non deve essere demonizzata *a priori*, ma presenta molte controindicazioni, perché da molti attenti operatori viene fatto rilevare che l'utilizzo dell'agente sotto copertura, proprio nei reati di corruzione ha delle controindicazioni perché tende ad intervenire

Sia sul piano investigativo, infatti, sia sul piano processuale che giurisprudenziale, esiste un consolidato (formatosi nel nostro Paese nella lotta al terrorismo e nella lotta alla mafia) che può essere trasferito

perché voglio riprendere un passaggio della sua replica. Vede, signor Ministro, questa norma, indipendentemente dall'emendamento, disegna e individua in maniera chiara come il Governo, nell'agire nella materia specifica, abbia avuto

Sostanzialmente, nel dover aggredire un fenomeno che non era casuale ed episodico (perché episodico e casuale è quel fenomeno che si ripete con riferimento a situazioni diverse), ma avendo a cuore i sistemi corruttivi che spesso si accompagnano alle grandi opere, il Governo ha pensato di inserire la legislazione premiale. Questo risulta in maniera evidente dal testo, che in parte ripete la formulazione della legislazione premiale in tema di terrorismo e di criminalità organizzata, ma che sostanzialmente punta ad evitare che l'azione delittuosa venga portata ad ulteriori conseguenze: evidentemente ciò non riguarda quel reato istantaneo che è la corruzione o la concussione, nonostante le acrobazie della Cassazione.

il relatore, non può essere considerato in termini assoluti, ma in termini relativi, rispetto al fatto concreto oggetto della fattispecie astratta. Ciò equivale a dire, signor Ministro, che nell'eventualità in cui il soggetto corruttore, attraverso le sue propalazioni, fa ottenere il sequestro della somma versata, magari indicando il conto estero su cui l'ha versata, sarà veramente difficile negare a quel corruttore la particolare circostanza attenuante che oggi prevediamo, perché sicuramente assicura il sequestro della somma e la sua condotta, in assoluto non efficace, è sicuramente efficace rispetto alla singola fattispecie. Ho ascoltando il senatore Lumia, in una ricostruzione storica del passato, e per la verità sono rimasto fortemente perplesso, perché che io ricordi, nel 1992, all'epoca di Tangentopoli poche furono le condanne per corruzione, ma davvero tante furono quelle per concussione e anzi - se lo vogliamo dire fino in fondo veniva favorito un dichiarare che puntasse verso la concussione, perché era il sistema e il modo per evitare la ricaduta, sotto il profilo della sanzione penale, che era propria della concussione.

Allora, signor Ministro, se questo è vero - e credo sulla base dell'esperienza pregressa possa essere difficilmente smentibile - vediamo come queste norme vanno a concatenarsi l'una con l'altra.

probabilmente non si riuscirà a dimostrare la concussione per costrizione, ma si dimostrerà la concussione per induzione

esame. Ciò vuole dire, signor Ministro, che l'errore di fondo di questo disegno di legge, ovvero aver immaginato una legislazione unica per i diversi tipi di corruzione, invece che immaginare una corruzione (e similari) - reato contro la pubblica amministrazione e una corruzione (e similari) - reato contro l'economia nazionale, porterà nella realtà a non vedere mai il corruttore in carcere. E questo sia perché riuscirà in qualche modo a convincere dell'esistenza della concussione per costrizione sia perché,

Credo che questo aumento di pena da un terzo a due terzi, destinato a valere per tutti i corruttori, sia davvero un fuor d'opera e non sia uno strumento utile a bloccare la corruzione. Che necessità ha il corruttore di accedere a quello che voi avete immaginato essere il patteggiamento condizionato, la restituzione del denaro per accedere al patteggiamento, se in ragione di questa norma, essendo sufficiente assicurare il sequestro del provento del reato, sfuggirà comunque al carcere avendo una diminuzione di pena di gran lunga maggiore rispetto a quella prevista in astratto dal patteggiamento?

di senso giuridico o molto lontane dalla pratica giudiziaria di questi ultimi anni. Il provvedimento andrà come andrà alla Camera,

Alla Camera potete ancora cambiare questo testo, potete ancora immaginare un sistema di contrasto alla grande corruzione più efficiente di quello che avete previsto e, ove mai dalla Camera dovesse provenire un testo in tal senso,

a contrastarlo nel rispetto dei principi generali del nostro ordinamento, nel rispetto delle garanzie costituzionali di tutti i cittadini.

soglie minime della pena perché non compatibili con i trattamenti premiali. Poi però ci si lamenta delle circostanze attenuanti che rendono queste pene minime compatibili con i trattamenti premiali. Mi rendo conto della difficoltà di argomentare su due versanti del tutto opposti pretendendo di fare opposizione su circostanze rispetto alle quali una scelta andrebbe fatta in una direzione o nell'altra. credo sia impensabile offrire all'Aula opinioni contrarie - ripeto - rispetto a norme che oltretutto sono funzionali a risolvere quei problemi di adattabilità delle pene minime a situazioni che siano altrettanto minime. Con questa premessa, credo intanto che questa norma sia funzionale, come dicevo nel mio precedente intervento, a determinare quell'incremento per le indagini che sfugge con riferimento alla punibilità dell'indebitamente indotto. Quindi è una norma funzionale anche a risolvere questo problema, lo dicevo allorquando esponevo le motivazioni della mia contrarietà ad emendamenti volti a sopprimere il secondo comma dell'articolo 319-*quater*. Questa norma però è funzionale anche a risolvere il problema, come dicevo poc'anzi, di soglie edittali ritenute troppo elevate; ossia chi vorrà fruire di un trattamento conforme, o per meglio dire compatibile con le misure premiali, sa in anticipo che c'è la strada di un contributo fattivo e funzionale in maniera efficace a consentire l'incremento del patrimonio conoscitivo del pubblico ministero, quindi il sistema su questo versante si presenta razionale. Ci sono i riti alternativi, le circostanze attenuanti generiche e, in aggiunta, l'attenuante di una collaborazione che consente a chi sia stato individuato non soltanto di contribuire efficacemente alle indagini, ma tra l'altro di avere un trattamento sanzionatorio conforme a quella che potrebbe essere una misura premiale. C'è da dire poi che si lamenta addirittura l'eccessività della riduzione della sanzione, quindi la la contraddittorietà si manifesta anche su questo ulteriore versante, allorquando si sostiene che è eccessivo ridurre la pena fino a due terzi. C'è da osservare, e l'osservazione è solo di natura tecnica, che l'attenuante è determinata con riferimento al minimo «da un terzo», cioè non si può scendere al di sotto del terzo, e con riferimento al massimo non oltre i «due terzi»; poi però nello spazio intermedio tra un terzo e due terzi il giudice potrà dettagliare la riduzione del trattamento sanzionatorio all'importanza, all'efficacia ed alla proficuità della collaborazione, come anche alla gravità del fatto, che rimane, a a prescindere dalla collaborazione. La norma quindi non è che dica che la pena è ridotta di due terzi, in modo che si possa dire che la riduzione è talmente imponente da imporre tra l'altro una riduzione obbligatoria al giudice, il minimo della riduzione che andava previsto è riferibile alla categoria delle circostanze comuni e ad effetto comune: «da un terzo», il massimo della riduzione di queste circostanze, ma poi spazia fino ai «due terzi», consentendo al giudice una determinazione in concreto corrispondente all'effettiva gravità del fatto, a prescindere dalla collaborazione.

chi ha la capacità di ragionare si rende conto che il ragionamento del presidente Palma era corretto anche sotto il profilo squisitamente tecnico. Per rispondere al relatore, senatore D'Ascola, dico semplicemente che l'adattabilità delle pene minime va immaginata nella determinazione delle pene minime, non attraverso un sistema di riduzione delle pene minime per effetto di un comportamento del soggetto imputato di questo reato nel corso del procedimento. quindi che i giudici debbano fare il loro lavoro, debbano individuare gli elementi di prova ed eventualmente sequestrare le somme, ma che non possano affidarsi, come per il passato è stato fatto, a chi va negli uffici di procura e, per evitare per sé la carcerazione, accusava gli altri. Sulla base di questo ragionamento, non posso che ritirare la firma dall'emendamento 1.342 ed al più ritengo di dovermi

nell'ottica del bilanciamento del potere sanzionatorio dello Stato, che deve comunque essere esercitato, al Movimento 5 Stelle sembra esagerata una riduzione che possa arrivare a due terzi della pena,

Pertanto, la posizione del Movimento 5 Stelle su questo emendamento sarà motivatamente contraria.

forzando un po' la lettura della *ratio* del provvedimento nel suo insieme - il presidente Palma, dall'aver messo al centro della nostra attenzione attenzione la «corruzione di nuovo conio», o meglio quella che si è sviluppata attorno alle grandi opere, legata alla costruzione di reti che hanno una una solidità e una diffusione consistenti. Essa deriva semplicemente dall'assunzione, all'interno del nostro ordinamento, compatibilmente con l'obbligatorietà dell'azione penale, di

sospetti dal punto di vista dell'adesione ai principi dello Stato di diritto, nei quali però non esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, prevedono nella prassi forme di incentivo alla collaborazione con chi esercita l'azione penale che vanno ben oltre la proposta contenuta nell'emendamento il presidente Palma ha posto incidentalmente un'altra questione, evidenziando che non abbiamo affrontato l'evoluzione del fenomeno corruttivo o forse l'abbiamo affrontata forzando l'impianto precedente, in questo modo snaturandolo. Ritengo non sia così. Ritengo che la flessibilità che ormai ha assunto il sistema, con l'introduzione del reato di induzione e con i meccanismi premiali, consenta di tener conto di questa evoluzione. Tuttavia, voglio dirlo perché non vorrei

tenendo insieme una serie di strumenti, che credo debbano essere messi tutti in relazione. Mi riferisco all'ipotesi di reato di corruzione tra privati, di cui stiamo attendendo una prima applicazione e il relativo consolidamento della giurisprudenza,

Io credo che, se si facesse una discussione che tiene insieme questi elementi, si affronterebbe seriamente il sistema. Nelle condizioni date e sulla base dell'impianto tradizionale, io credo però che abbiamo introdotto alcuni elementi che consentono di tener conto di questa evoluzione, che è stata rapida e lo sarà ancora di più nei prossimi anni, perché sappiamo che i fenomeni criminali spesso evolvono molto più rapidamente della legislazione. Se quel tipo di fenomeni li vogliamo leggere e li vogliamo interpretare,

per mettere in discussione il lavoro fatto fin qua, ma semmai per proporre un altro terreno di lavoro, che non comprometta l'approvazione rapida di questo provvedimento, ma che consenta di aprire un altro campo di lavoro e di individuare nuovi strumenti.

sarebbe potuto aprire uno spazio per una diversa collaborazione anche da parte dell'opposizione, con una valutazione seria, proprio in base ai principi che lei ha affermato e di quello che stiamo votando, anche sotto il profilo delle pene. Io sono convinto di quello che lei ha detto e, per questa ragione, sono intervenuto per ringraziarla, augurandomi che queste cose si dicano e si facciano per realizzare un accordo e un'unità e non nel momento in cui si tratta soltanto di acquisire dei consensi, come il mio, che poi non danno risultati.

questo emendamento, che ho già illustrato precedentemente, è volto a richiamare l'attenzione sul fatto che la corruzione a volte è anche generata da atteggiamenti dei pubblici uffici, che non fanno ciò che devono oppure lo fanno in tempi inenarrabili. Naturalmente una dazione può accorciare i tempi. E qui non si tratta di avere o non avere pazienza; a volte ci sono aziende che falliscono,

importante che ci sia questa controparte. Vorrei ricordare che il fenomeno non può essere ridotto alla mera repressione o al mero aumento delle pene perché, a proposito di statistiche sulla corruzione, ogni giorno siamo martellati dai *media* (90 per cento, 102 per cento), ma - ripeto - è corruzione percepita. La domanda principale che viene fatta

ricevuto la proposta di prendere dei soldi e in cambio fare qualcosa di contrario ai suoi doveri: questa è una statistica seria e dà

nel frattempo non si possono essere esercitare i propri diritti. Evidentemente ci sono ancora troppi casi per cui si pensa che denunciare non serve a niente, perché c'è il rischio che chi denuncia finisca ancora più nei guai di colui che viene denunciato, perché a denunciare certi personaggi potenti c'è il rischio di finire male. È in questa direzione, semmai, che bisognerebbe agire. A questo tendeva il mio emendamento. Tuttavia, di fronte al parere contrario del relatore e al timore che non sia correttamente inserito dal punto di vista tecnico, lo ritiro.

perché il Ministro ha capito, nel dibattito che si è svolto in quest'Aula, che va riscritto il Libro II del codice penale,

di una valutazione complessiva che non può prescindere da una riconsiderazione del Titolo

ma essendo stato costretto per anni ad interessarmi dell'economia per gli effetti sulla giustizia, noi dobbiamo oggi preoccuparci anche dei comportamenti che interessano la giustizia ma che hanno un'influenza sull'economia nazionale. nazionale. Credo sia giunto il momento di avere un Capo del codice penale dedicato ai delitti contro l'economia nazionale.

si è ridotta di gran lunga l'efficacia di deterrenza delle norme sui delitti contro il patrimonio che incidono sull'economia nazionale. Dall'altro lato, noi assistiamo a un sistema del nostro Paese che è organizzato

sostenendo l'accusa in uno dei procedimenti di Mani pulite, sostenni che era necessario addivenire a una riscrittura delle regole degli appalti, in particolare sulle revisioni in corso d'opera. Esistono due possibilità di corruzione: o la revisione in corso d'opera la sottoponiamo alle stesse regole che disciplinano le gare d'appalto,

l'intervento di autorità che possa evitare che si verifichino fatti di rilevanza penale.

che era il centro di elaborazione culturale e politica del vecchio Partito Comunista. Nel Centro per la riforma dello Stato si discuteva e si sosteneva che la nostra Costituzione è fondata sul sistema dei controlli. È solo sul sistema dei controlli che si fonda la nostra democrazia. Ma questo sistema dei controlli deve essere rapportato alle sanzioni e alle norme incriminatrici dal punto di vista penale. penale. Come può andare avanti un sistema economico se è aggredito dalle norme che riguardano i diritti contro il patrimonio, che non hanno più alcuna efficacia di deterrenza?

probabilmente la situazione economica di alcune famiglie porta anche a queste follie. Ma guardiamo alla realtà economica del nostro Paese.

ci porta a dire che forse abbiamo ragionato diversamente in Commissione e nessuno ci ha seguito.

in cui è espressa l'indicazione di applicare le norme dal comma 15 al comma 36 della legge Severino che riguardano la trasparenza.

perché solo allora noi potremo dire di aver fatto il nostro dovere, cioè di aver contribuito non a mettere in galera le persone, dato che non serve, ma a riformare un sistema penale in coerenza con le nostre finalità e, allo stesso tempo, ad offrire un contributo serio all'economia nazionale.

Presidente, la riformulazione suggerita dal Governo, che io non ritengo di accettare, per la verità non è di poco conto. Sostanzialmente si chiede di eliminare il termine «modificato». Ora, se il Governo è convinto Governo è convinto di intervenire per operare una giusta distinzione tra i reati di corruzione che vanno ad incidere sull'economia

ed esprimere un parere favorevole su questo ordine del giorno, che chiude le porte ad ogni modifica, mi domando che cosa significhi. Perché mai il Governo accetta l'invito di integrare il testo e non già di modificarlo? Che cosa significa integrare?

3.0.304, 5.0.302, 7.0.301, 7.0.302, 7.0.303, 7.0.304, 7.0.305, 7.0.306,

11.0.301, 11.0.302 e 11.0.309 che recano disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge in esame. Risultano altresì inammissibili 1'emendamento 4.0.303, in quanto privo di portata modificativa, nonché le proposte 1.0.305, 1.0.306, 1.0.307, 1.0.308,

«(Operazioni sotto copertura)». Le parole: «e agente provocatore» sono da ritenersi cassate perché non c'è la disciplina dell'agente provocatore in questo emendamento del quale stiamo

Nel suo intervento - che condivido - il collega Malan ha citato, senza ovviamente rivelare la fonte, la Commissione costituita presso il Ministero della funzione pubblica dal ministro Patroni Griffi nel 2012,

Tutto questo non portava a quella cifra di appena 100 milioni in tre anni, ma portava alla cifra di oltre 300 miliardi in tre anni. La proporzione (o la sproporzione) è sotto gli occhi di tutti. Cari colleghi, voi non volete intervenire su questo sperpero di denaro pubblico, sulla vischiosità, sulla farraginosità, sulla burocrazia inutile e sui 1000 passaggi. Voi non sapete che un cittadino che deve avviare una attività

migliaia di agenti pubblici distolti dall'attenzione dei fatti criminali e di terrorismo che stanno toccando Paesi vicini a noi: dalla Francia, al Belgio, all'Olanda, alla Tunisia.

Le vere leggi che dobbiamo fare sono quelle di interesse sociale: sono quei ponti che vengono fatti senza strade di accesso. Sono quelle strade che finiscono nei fiumi che non hanno più ponti. Sono quelle opere che vediamo in certe trasmissioni televisive (come «Striscia la notizia»), che a volte fanno delle indagini e dei

di tutto e di più. Certamente parliamo di un reato di grande interesse sociale e qui, nel tempio della democrazia, sento mercanti che bisognerebbe cacciare: ma faccio finta di non sentire perché non sono Cristo e ovviamente non ho la frusta per cacciarli.

in fin dei conti esso prevede un'ipotesi aggravata di concussione, ove la concussione venga posta in essere da un appartenente all'ordine giudiziario. Mi permetto di ricordare a tutti che si configura un'ipotesi più grave ed autonoma di corruzione ogni qualvolta quella corruzione viene posta in essere da un appartenente all'ordine giudiziario. Poiché credo che nel nostro codice vi debba essere una simmetria, così come prevediamo un'ipotesi aggravata (la corruzione in atti giudiziari) in quanto commessa da un appartenente all'ordine giudiziario, non credo che si possa liquidare così facilmente, al di là della formulazione, un emendamento che tende ad instaurare una figura simile con riferimento al più grave reato di concussione. Se il relatore ed il Governo sono d'accordo, avviando alla conclusione, accantonare questo emendamento, anche per consentire, se del caso, delle riformulazioni e per approfondire la materia, perché oggettivamente vi sarebbe un vuoto.

da chi amministra la giustizia, dall'imbuto finale che deve giudicare e che agisce per fini suoi personali?

Presidente, l'aumento della metà porta ad una pena minima di nove anni e ad una pena massima di diciotto Il che vuol dire - e lei me lo insegna - che anche con le attenuanti generiche si sta sempre al di sopra dei cinque anni, e con i cinque anni scatta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

che è una pena accessoria.

Insomma, mi dovete spiegare una cosa: per quale ragione, se la corruzione riguarda un giudice, la pena viene aumentata, perché diversa è la pena per la corruzione in atti giudiziari rispetto alla corruzione normale, e invece per la concussione la pena deve essere assolutamente uguale, anche quando la concussione viene fatta dal giudice? Non riesco a comprendere la ragione per la quale aggraviamo il reato di corruzione e non aggraviamo il più grave reato di concussione, quando sostanzialmente la vita di una persona è esattamente nelle mani di quel giudice che va a chiedere i soldi. È per questo che avevo chiesto un accantonamento. Ora lasciamo perdere la questione dell'interdizione perpetua; qui la cosa interessante è che c'è un aumento di pena Allora voglio dire una cosa: ma davvero voi ritenete che non possa esistere un giudice concussore, pur esistendo un giudice corrotto? Ma che legislazione stiamo facendo? Quindi, non essendo possibile un accantonamento, mi auguro che il senatore Barani voglia togliere almeno l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché questa parte è superata dalla disciplina generale. Se restano le parole «Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà», il Gruppo di Forza Italia voterà a favore.

"Il link apre una nuova finestra") che ho presentato giovedì scorso, all'indirizzo del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia, che io credo presenti caratteri di indubbia urgenza ed importanza. So bene che qualcuno, visto l'andazzo registrato in questa legislatura sui tempi di risposta, potrebbe sorprendersi della mia sollecitazione, ma i temi in questione impongono uno sforzo ed un'attenzione straordinaria. Mi riferisco alle pesanti e assurde ricadute di natura economica che si stanno determinando sulle persone con disabilità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole per il calcolo dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Le chiedo pertanto di sollecitare, con ogni mezzo, l'Esecutivo a fornire il prima possibile una risposta a questo atto di sindacato ispettivo e, comunque, in tempi utili a garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la dichiarazione dei redditi, chiarendoci soprattutto la posizione che il Governo intende assumere su tale questione, anche alla luce delle tre diverse sentenze del TAR Lazio, che hanno stroncato, senza appello - oserei dire - queste nuove disposizioni. La prego di intervenire e di sollecitare il Governo perché c'è un mondo, quello, purtroppo, dei portatori di disabilità, che è in apprensione e in confusione perché non sa come comportarsi in vista della dichiarazione dei redditi.